L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, il provvedimento in esame costringe tutti a rendersi conto della necessità, ancora più evidente, di una profonda riforma dell'università; una riforma che abbia requisiti di organicità e completezza...

una struttura piramidale della docenza, che non è più tanto tale perché ha una base troppo ristretta ed un vertice troppo largo; una mancanza di finanziamenti alla ricerca adeguata alle necessità del momento e, a voler essere critici, anche la necessità di nuovi tipi di vaglio sul finanziamento alla ricerca, per fare in modo che i finanziamenti, pur scarsi e sempre insufficienti, possano essere indirizzati verso le ricerche più significative. Di fronte a queste necessità, il provvedimento offre scarse risposte. È già stato osservato da molti colleghi che i provvedimenti che portano il cognome del ministro Gelmini, sulla scuola inferiore e quello in esame, soggiacciono in una maniera schiacciante all'imperio della legge n. 133 che imprime a tutta la gestione del finanziamento pubblico la logica di un taglio pervasivo, incisivo e in qualche caso rovinoso. Mentre, però, il provvedimento sulla scuola inferiore ha avuto quasi esclusivamente questo carattere, con una cosmesi di restaurazione dei valori puramente conclamata, bisogna riconoscere che nel provvedimento in esame il Governo ha fatto lo sforzo di considerare con maggiore attenzione per lo meno alcune questioni. Ovviamente l'Assemblea è sovrana e decide secondo il proprio libero intendimento. Io credo che sia difficile sottrarsi alla tentazione di pensare che la maggioranza abbia avuto un atto di resipiscenza operosa, seguito ad una certa comprensione di ciò che i movimenti degli studenti, dei ricercatori, dei professori e delle famiglie hanno chiesto in maniera vigorosa, pacifica,

tributo alla maggioranza il riconoscimento del fatto che essa ha in un certo senso accolto qualche motivo della protesta sociale, ma ritengo che la causa fondamentale di tale resipiscenza operosa sia proprio da individuare nella capacità di convincimento che i movimenti hanno esercitato. Tuttavia, all'interno di questo provvedimento permangono luci ed ombre. Parto dagli aspetti meno negativi. A mio avviso, sono meno negativi il riconoscimento che bisogna ampliare il *turnover* dal 20, come era stato promesso all'inizio della legge finanziaria, al 50 per cento: si riapre l'orizzonte.

nei futuri concorsi, perché, in fondo, in questa maniera si accetta in qualche misura, secondo me insufficiente, il criterio secondo il quale occorre riallargare la base della piramide della docenza e della ricerca e provare a rastremare un po' i vertici. Tra i motivi che mi fanno giudicare non del tutto negativo il provvedimento c'è anche una certa, modesta, riapertura del finanziamento.

è soltanto provvisorio e temporaneo: basta che le università si rimettano in moto e tale confine verrà rapidamente varcato e quasi tutte le università diventeranno meno virtuose. sui criteri del reclutamento il collega Livi Bacci ha detto una cosa giusta: è del tutto inesplicabile fissare nelle commissioni di concorso la sola presenza di professori ordinari; non ha senso, per mille motivi, che si possono sintetizzare così: i professori associati hanno diritto di avere per lo meno un loro collega nelle commissioni di concorso ed i ricercatori lo stesso, non per una questione corporativa, corporativa, ma di comunità scientifica, di adesione ai nuovi aspetti della ricerca su cui le forze giovani sono probabilmente più in contatto. Trovo anche che abbia qualche carattere di puerilità la questione dell'obbligo di pubblicazione. È un'esigenza sacrosanta: i professori non possono fare i professori se non pubblicano qualcosa. Però, vedete, applicando alla stretta tale criterio uno dei più celebri autori dell'economia politica del secolo precedente, Piero Sraffa, autore di un solo libretto di 60 pagine, intitolato: «Produzione di merci a mezzo di merci»,

Insomma, c'è una questione di misura della qualità. Forse bisognerebbe allora insistere non tanto sul limite temporale dei due-tre anni e sulla quantità di pubblicazioni, quanto sulla possibilità di giudicare invece la qualità, che è cosa molto più difficile e molto più ardua e che richiede Un altro elemento negativo, e qui ritorno il provvedimento soggiace in maniera irrimediabile alla potenza della legge finanziaria.

può anche darsi benissimo che i finanziamenti privati possano dare ristoro ad un mondo esausto e magari invogliare persino certe direzioni di ricerca, immagino immagino soprattutto quelle che hanno a portata di mano nel giro di breve tempo un qualche risultato economico; bisogna vegliare sulla cosa. Sono contento che la maggioranza abbia accolto il suggerimento intrinseco in un ordine del giorno che è stato accolto e cerca di porre rimedio alla possibilità di alienazione dei beni universitari una volta che arrivino le fondazioni private ad esercitarvi un qualche controllo. Ma vi è anche una questione di libertà della ricerca. infatti, immaginare che la ricerca possa essere indirizzata da fonti private verso esiti di interesse privatistico è molto più difficile immaginare che la libertà della ricerca disinteressata possa essere salvaguardata. Mi riservo un'altra occasione per cantare le lodi della ricerca disinteressata, mi limito oggi ad accennare brevemente che il campo del sapere è ricco di varianti, di cunicoli, di piccoli corridoi, di stanze segrete, di campi poco frequentati, in cui vale anche l'applicazione di una sola mente su un solo problema.

Vi faccio solo un esempio: io ho una bravissima allieva, dottore di ricerca, che ha pubblicato un libro, che ha insegnato all'estero, che non è ricercatrice perché non può esserlo, perché non potrà vincere un concorso, quale tiene un corso di 72 ore con 200 studenti all'università di Firenze e viene pagata 3 euro a lezione. Tiene un intero corso universitario e alla fine il pagamento del suo corso è inferiore a 300 euro, e questi 300 euro gli vengono pagati in due rate, 150 all'inizio e 150 alla fine. Voi pensate che si possa gestire l'università in questo modo? A Firenze nella mia facoltà gli strutturati sono 140, i precari sono 241: giudicate voi.

è un fatto che molti atenei hanno prodotto voragini di bilancio. La riforma del cosiddetto "3+2" ha moltiplicato le cattedre: il numero dei docenti supera in alcuni corsi il numero degli studenti iscritti, addirittura vi sono corsi universitari con un solo iscritto e sedi distaccate inutili. È una situazione ai limiti dell'incredibile, che impone interventi decisi e mirati. Di certo, come Lega Nord, faremo da cani da guardia contro sprechi, baronati e clan familiari. Ma soprattutto, come Lega Nord, non possiamo non denunciare la situazione paradossale che vede le più produttive università del Nord penalizzate finanziariamente, mentre quelle del Sud ricevono più soldi di quelli che le spetterebbero.

E questo - trattandosi in molti casi di formazione altamente strategica in quanto connessa col mondo della ricerca e dello sviluppo, con tutte le ricadute del caso in termini di conoscenza scientifica e di applicazioni in campo economico - è decisamente grave. Nel 2007 le sette università lombarde finanziate dallo Stato hanno ricevuto in totale 832 milioni di euro, quando invece, sulla base dei requisiti di efficienza in passato elaborati dal Ministero competente ma mai applicati, avrebbero dovuto riceverne 935. Per gli atenei della Lombardia manca quindi all'appello una media dell'11 per cento dei fondi; un ammanco che nel caso specifico del Politecnico di Milano raggiunge il 24 per cento, risultante dall'acquisizione di 192 milioni anziché dei 235 dovuti. di peggio: l'università di Bergamo doveva ricevere 47 milioni, ma in realtà ne sono arrivati 32, cioè circa il 30 per cento Opposta è la situazione della Sicilia, le cui università hanno avuto, lo scorso anno, una media del 20 per cento in più del dovuto, per l'esattezza 622 milioni anziché 496.

La Campania guadagna un buon 7 per cento, con una punta del 13 per cento per la Seconda università di Napoli, che ha avuto 134 milioni in luogo di 116. Opposta la situazione delle università del Piemonte, sottofinanziate in media del 16

(ma con l'ateneo di Udine sottofinanziato di 12 milioni, corrispondenti a un meno 17 per cento) e la Liguria, che all'università di Genova ha visto arrivare il 12 per Certamente anche al Sud non mancano Regioni le cui università sono sottofinanziate, come Calabria e Abruzzo, ferme in entrambe sul meno 15-16 per cento. Tuttavia, è evidente che a fare le spese della situazione sono principalmente le facoltà del Nord, quelle che costituiscono il principale motore del Paese. Complessivamente, le università di Sicilia e Lazio risultano sovrafinanziate rispettivamente di 125 e 85 milioni di euro; l'opposto del Nord, che vede gli atenei lombardi sottofinanziati per 93 milioni di euro, quelli piemontesi per 63 milioni, e quelli veneti per 47 milioni. Il primo tentativo di elaborare criteri di valutazione a cui agganciare i finanziamenti risale a metà degli anni Novanta. Nel 2004 viene fissato il cosiddetto modello di ripartizione del fondo per le università, un modello che tiene conto, per ciascun ateneo, del numero di iscritti, del totale degli esami superati e dei laureati, dei risultati della ricerca. Tali criteri, studiati a tavolino, sono però rimasti per lo più lettera morta: i finanziamenti sono stati erogati secondo quote storiche di spesa. In sostanza, ciascun ateneo, efficiente o meno che fosse, ha continuato a ricever le stesse somme, premiando così le università sprecone, prive di incentivi a cambiare rotta. Si calcola che, tra il 2003 e il 2007, il sistema universitario italiano abbia ricevuto dallo Stato quasi 34 miliardi di euro, ma di questi appena 540 milioni sono andati realmente alle università migliori in termini di efficienza, qualità e assenza di sprechi. Anche il tentativo nel 2007 dell'Esecutivo di centrosinistra di elargire 400 milioni di euro, cioè il 5 per cento dei finanziamenti statali per gli atenei, indirizzandoli agli istituti di maggiore qualità, è fallito. Ora, con l'articolo 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge n. 180 del 2008, succede qualcosa che per l'Italia anche qualche rappresentante dell'opposizione non ha potuto che definire rivoluzionario. Il suddetto articolo che: «A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario (...) e del fondo straordinario (...), con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione: la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; *b)* la qualità della ricerca scientifica; *c)* la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche». Tradotto in soldoni, ciò vuol dire che, da subito, 500 milioni di euro saranno finalmente destinati a premiare le università più virtuose. Entro il 2011 gli stanziamenti destinati agli atenei meritevoli dovrebbero salire a 1,8 miliardi di euro, cifra che equivale al 30 per cento del finanziamento pubblico complessivo al sistema universitario, attualmente stimato sui 7,4 miliardi di euro, e che - è vero - in conseguenza dell'attuale crisi economica fra 3 anni potrebbe scendere a 6 miliardi. Ma i fondi finalmente andranno a chi li merita. Tornando al decreto in discussione, oltre ai 500 milioni da distribuire con criteri meritocratici, ci sono 135 milioni affinché possano avere una borsa di studio tutti i circa 180.000 ragazzi che ne hanno diritto (fino a oggi riuscivano a ottenerla solo 140.000 studenti) e 65 milioni per alloggi e residenze universitarie. Sono inoltre previsti 4.000 posti in più per i ricercatori, grazie a un investimento di 150 milioni, con l'obiettivo di diminuire l'età media dei docenti. Almeno il 60 per cento delle assunzioni dovranno essere riservate a nuovi ricercatori. Gli atenei che non tratterranno i docenti con più di 70 anni potranno raddoppiare il numero dei posti per ricercatori. tutti interventi che la Lega Nord apprezza, perché non chiediamo privilegi, ma di mettere - in base a quanto spetta - i diversi territori in condizioni di reggere la competizione internazionale. La strada - nell'ottica della concretizzazione del federalismo fiscale - è quella della meritocrazia, dell'efficienza e della lotta agli sprechi (sui parametri da utilizzare avremo abbondantemente modo di confrontarci). Concludo dichiarando il voto favorevole della Lega Nord, che considera fondamentale finanziare l'università secondo criteri e parametri ben definiti e vincolati alla riqualificazione e al controllo della spesa e a precisi obiettivi di rilancio, finalizzati all'incentivazione del merito e dei livelli qualitativi della formazione e della ricerca. Finanziamenti che possano valorizzare la posizione dei giovani più meritevoli e favorirne l'attività, in un contesto che preveda l'attivazione di un adeguato sistema di valutazione e verifica dei risultati. Non può esserci autonomia senza responsabilità.

un professore universitario prestato alla politica, mi sento onorato di frequentare da qualche mese quest'Aula, da trent'anni frequento

e poi una speranza. I modi in cui nel Paese si è aperto il dibattito sull'università sono motivo di seria preoccupazione e questo decreto, al di là delle sue motivazioni, che in parte - come dirò condividiamo, si è prestato ad essere di fatto causa ed effetto di questi modi e dello spostamento dell'attenzione su questioni non sostanziali. La crisi dell'università non può essere affrontata a partire dai suoi sintomi più superficiali, anzi fare questo può essere addirittura controproducente, si tratta infatti di una crisi strutturale dell'università, una crisi che dipende non non da isolati casi di corrompimento della vita accademica, ma dai grandi cambiamenti sociali indotti dalla globalizzazione e dai cambiamenti che riguardano la produzione e l'organizzazione dei saperi oggi. Mai nella storia umana come in questi ultimi venti anni si erano prodotti così radicali e così rapidi cambiamenti nella società e nella conoscenza. È proprio questo che ci impone di ripensare alla radice, con coraggio, con coscienza e con conoscenza il sistema universitario: dobbiamo riattualizzare le sue finalità (la formazione e la ricerca), dobbiamo riconsiderare il complesso delle funzioni decisionali, la composizione dei vari organi, il loro ruolo, le loro responsabilità nella programmazione e nella gestione delle risorse, ma proprio a questo scopo la politica e il Parlamento devono e possono oggi tornare ad essere il luogo di un grande progetto ed è ancora proprio per questo che l'università deve essere concepita come la risorsa da cui attingere idee. Ieri osservava opportunamente e vigorosamente il senatore, professor Livi Bacci, che l'università italiana non è da punire, non è da umiliare o addirittura da buttare. Rispetto ai cambiamenti che hanno investito la società è indubbio che il ruolo dell'università e la funzione sociale a cui deve corrispondere abbiano subito bruschi rivolgimenti: da luogo di formazione di *élite*, l'università si è trovata a fare fronte ad una domanda di formazione straordinariamente aumentata. Oggi l'80 per cento dei diplomati accede all'università, La nostra università negli ultimi dieci anni ha aumentato le immatricolazioni, nonostante una diminuzione del numero dei giovani tra i 18 e i 20 anni, e ha più che raddoppiato il numero dei laureati in sette anni: da 140.000 nel 2000, oggi sono 300.000. che se ciò significa da un lato democratizzazione della cultura e dell'accesso all'alta cultura, dall'altro implica anche una moltiplicazione e una profonda diversificazione delle richieste di formazione. La sfida sarà quella, come in ogni Paese democratico e sviluppato, di coniugare sapientemente la democratizzazione della cultura con la valorizzazione del merito e dell'eccellenza; ma all'esame affronta con misure di urgenza una materia che dovrebbe invece essere oggetto di progettazione approfondita e condivisa, senza prescindere da una visione di insieme dell'esigenza dell'intero sistema. È controproducente che mutamenti di tale portata possano essere definiti frettolosamente, sulla base di mere considerazioni di spesa, tramite un decreto-legge che, ancora una volta, esautora il Parlamento delle sue prerogative e ricchezze di contributo possibili. Lo abbiamo sperimentato in queste poche settimane, purtroppo in tempi rapidi, nelle interessanti discussioni in 7a Commissione, grazie ai contributi di tutti, maggioranza e minoranza, in particolare grazie al lavoro del presidente Possa e del relatore Valditara. Sarebbe stato e sarebbe per questo importante - questa è la speranza - trasferire quel metodo, Il decreto, così concepito, ha avuto conseguenze comunque negative. Il metodo per affrontare il problema è diventato esso stesso il problema; nel merito il decreto contiene indicazioni e obiettivi generali che possiamo sostanzialmente condividere, ma corrisponde nell'insieme ad una inutile dilazione di provvedimenti più importanti e non sposta la pesante ipoteca della legge n. 133, che grava su di lui. Il decreto è l'effetto collaterale di una finanziaria che taglia radicalmente gli investimenti sulla formazione e sulla ricerca. Certo, esso introduce qualche rimedio per il prossimo anno, ma il taglio di un miliardo e mezzo di euro, previsto dalla legge n. 133, permane come un macigno. Il decreto, dunque, come ha osservato anche il professor Decleva, presidente della Conferenza dei rettori, se non sostenuto da altre iniziative che modifichino i tagli dei trasferimenti nel 2010, sarà irrilevante nelle conseguenze che Nel provvedimento si intendono penalizzare gli atenei non virtuosi, quelli che superano il tetto del 90 per cento del proprio bilancio per coprire le spese di personale.

Inoltre, con i trasferimenti previsti nel 2010, anche il *turnover* del 50 per cento, che avrebbe comunque l'effetto meritorio di agevolare l'accesso al lavoro universitario di giovani ricercatori, non potrà essere applicato dalla quasi totalità delle università, perché tra un anno diventeranno non virtuose. I criteri proposti dal decreto per formare le commissioni dei concorsi, poi è l'oggetto più dibattuto, e anche male, purtroppo, sulla stampa - si affidano al metodo del semi sorteggio. Con l'intento di risolvere urgentemente i difetti del sistema vigente, il decreto introduce un metodo che già non aveva dato buona prova di sé in passato. Nessuno di noi ha paura del sorteggio, nessuno; avrebbe anche potuto essere più opportunamente totale, più radicale. Il problema è innanzi tutto, però, di non avere paura, piuttosto, della responsabilità, e per questo neanche dell'autonomia, il problema del reclutamento ha bisogno di un progetto complessivo, volto davvero e finalmente alla valorizzazione e all'incentivazione del merito e dell'eccellenza. Il mondo universitario è stanco dell'inerzia, è stanco del grigiore; lo sanno il professor Possa e il professor Valditara. Grigiore e inerzia nel nostro mondo universitario provocano solo involuzione, ma il mondo universitario è stanco anche di provvedimenti tampone che sono controproducenti. Abbiamo bisogno di un progetto di riforma radicale e sostanziale. La nostra contrarietà a questo decreto ha a che fare con il metodo, un decreto appunto, che ha il solo effetto di avere già rinviato ancora una volta la definizione di un disegno di legge. È a questo che noi stiamo già lavorando; a questo siamo interessati e chiediamo alla maggioranza di discutere rompendo ogni indugio. Questo è necessario, improcrastinabile e possibile. Nel merito, questo decreto rischia di produrre effetti contrari a quelli dichiarati. La manovra economica che lo ispira o lo condiziona, se non vi sarà un rapido cambiamento di rotta, rischia di coincidere con un sostanziale e pericoloso disimpegno dello Stato rispetto all'università. Per queste ragioni il Gruppo del Partito Democratico esprime un voto negativo su questo decreto proprio perché siamo impegnati e ci impegniamo nella costruzione di un progetto complessivo di riforma dell'università capace di portare gli atenei italiani a quell'eccellenza che è il vanto della tradizione plurisecolare del nostro Paese. Per questi ragioni il Partito Democratico esprimerà voto contrario a questo decreto.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori**,** è passato meno di un mese da quando in questa Aula l'approvazione di un decreto sulla scuola è stata presa a pretesto per scatenare una battaglia mediatica che aveva come tema la presunta volontà del centrodestra e del suo ministro Gelmini di mettere in ginocchio l'università italiana. Si protestava contro una riforma che non c'era e che, come dirò tra breve, non c'è. Cos'è successo in questo mese? Innanzitutto si è chiarito ancora meglio quanto sia profonda la crisi dell'università italiana; si è capito che questa crisi non dipende unicamente e nemmeno prioritariamente dai finanziamenti. È, invece, una crisi morale e di sprechi, una crisi di inaccettabili privilegi, una crisi di egoismi corporativi. Prendiamo un esempio emblematico: il caso dell'università di Siena. Si tratta certamente di un'università che nessuno può sospettare sia stata governata dal centrodestra e che si è risvegliata un bel mattino con circa 200 milioni di euro di debiti; un debito che si è consolidato nel tempo, che non dipende né dal Ministro Mussi né tantomeno dal ministro Gelmini e che non è nemmeno unicamente imputabile a questo o a quel rettore perché coinvolge responsabilità di controllo dei bilanci che devono essere accertate dagli organi competenti. Per questo il caso Siena consente discorsi non ideologici. In due giorni in quella università e all'unanimità per salvarla sono stati chiusi oltre 30 corsi di laurea giudicati inutili; le sedi distaccate sono state portate da cinque a due perché nelle altre c'era un numero di docenti superiore al numero degli studenti. I dipartimenti sono stati accorpati per evitare sprechi e privilegi baronali; é stato decretato il blocco delle assunzioni per adeguare il numero dei docenti al numero degli studenti. Si è varato, infine, un piano di dismissione degli immobili superflui per coprire il debito pregresso; il tutto per portare il bilancio in pareggio nel 2012. É stato fatto, cioè, senza nessuna imposizione del Governo, sulla base del buon senso e all'unanimità, quello che è stato contestato a questo Governo. Se si terrà fede a ciò che è stato dichiarato - e noi da parte nostra controlleremo che si tenga fede - Siena potrebbe diventare un caso emblematico per tutta l'università italiana. Così come, per molti versi, emblematico è il decreto-legge che oggi ci accingiamo ad approvare. La senatrice Garavaglia ha detto che non si tratta di una riforma. Diciamo allora che è il vagone di testa che dà la direzione ai convogli che seguiranno e che il Ministro ha descritto nelle linee guida per l'università, che ci ha fatto avere qualche giorno fa. Emblematica è anche la norma sui concorsi. Il collega Livi Bacci, che conosce l'università come forse nessun altro in questa Aula, ha affermato che non c'è sistema di concorso che non possa essere manipolato. È un modo per dire che nulla può sostituire la qualità etica delle persone. Ciò nondimeno, di fronte ad un sistema che anche di recente ha prodotto nepotismo, ha scoraggiato la mobilità, ha trasformato la logica di merito in una logica di avanzamento per anzianità, era doveroso dare un segno di discontinuità. E a volte gli emblemi servono quanto le riforme strutturali. Per quel che concerne i concorsi, lo possiamo oggi forse capire meglio di fronte allo spettacolo offerto dall'ultimo concorso in magistratura e alla prospettiva che vi sia chi possa arrivare a giudicare della libertà dei suoi simili attraverso un imbroglio. Quando queste cose accadono nell'università o nella magistratura,

Si temeva che la norma sui concorsi potesse essere edulcorata qui in Senato da pressioni corporative. In passato questo era accaduto. Questa volta no, per la volontà congiunta del Governo e dei Gruppi di maggioranza. Ed è, questo, un esempio virtuoso di quel *continuum* tra Governo e maggioranza che noi sosteniamo come una delle novità di questa legislatura e che a lei, senatrice Finocchiaro, tanto dispiace. Per il resto, con questo decreto-legge si afferma il criterio in base al quale i soldi debbono seguire il merito. Lo si fa stanziando 500 milioni di euro per le università virtuose e penalizzando, nelle assunzioni, gli atenei con bilanci critici. inoltre, si rafforza il diritto allo studio e, soprattutto, si svecchia una università nella quale, a causa di logiche corporative, i professori ordinari sarebbero presto diventati più numerosi dei ricercatori. Si inverte, cioè, quella piramide che la logica del privilegio aveva rovesciato, tornando alla fisiologia di ogni accademia. Il decreto-legge in Senato è stato ulteriormente arricchito con emendamenti che vanno nel senso di rafforzare ancora di più il merito e di consentire la valutazione. L'anagrafe dei docenti universitari, il divieto per chi non produce scientificamente di partecipare ai concorsi come commissario e di ricevere fondi di ricerca pubblici, sono altri atti concreti che il lavoro della maggioranza in Commissione consente oggi di mettere all'attivo di questo provvedimento. Non è la riforma, senatrice Garavaglia, ma è qualcosa che smentisce radicalmente l'accusa per la quale i tagli erano fini a se stessi. *(Applausi Non a caso, per andare avanti in questa stessa direzione, abbiamo voluto un'indagine conoscitiva sulle università italiane che chiarisse a tutto il Parlamento la situazione del loro bilanci, la realtà, oscura 5.500 corsi di laurea e lo sperpero causato da sedi nelle quali spesso i docenti sono più degli allievi. È qualcosa che smentisce le accuse infamanti che hanno ricoperto per un mese il Governo e il ministro Gelmini. *(Applausi di dialogo a quei ragazzi che avevano protestato, spesso in buona fede, ai quali offriamo fatti sui quali riflettere e non benevolenza a buon mercato. È, soprattutto, una risposta a quei tanti giovani che, per dirla con Prezzolini, non l'hanno bevuta. Ai tanti milioni che non sono scesi in piazza, ai centomila che hanno firmato la petizione della maggioranza silenziosa nella quale rivendicano il loro diritto di continuare a studiare. È una risposta a quanti all'università La Sapienza, proprio laddove la protesta è stata più forte, hanno votato per le liste indipendenti e di centro-destra, condannando la sinistra ad una sconfitta emblematica. *(Vivi,

Ci limitiamo a chiedere all'opposizione il rispetto per questi giovani, a non dimenticarli al primo stornir di corteo, così come noi rispettiamo chi protesta entro i confini della legge. E un'ultima considerazione me la deve, Presidente, e ho concluso. Ieri sera non è stata scritta una bella pagina nel rapporto tra maggioranza e opposizione. *(Prolungati Conosciamo la durezza della lotta e anche la necessità a volte di non fare sconti: l'abbiamo praticata nella scorsa legislatura. Ma sappiamo anche che la lotta politica, anche la più aspra, può e deve contemplare il *fair play*. Oggi, la maggioranza è al suo posto, più numerosa di ieri come è doveroso per una maggioranza che si rispetti e che si vuol far rispettare: nessun atto di eroismo. L'opposizione, oggi, non c'è: e questo segna la distanza tra una legittima e dura iniziativa politica e un prepotente dispetto che nasconde impotenza. *(Vivi, Onorevoli colleghi, il relatore, senatore Valditara, ha segnalato un errore materiale nella formulazione dell'emendamento 1.2010, preventivamente approvato dalla Commissione e quindi dall'Assemblea. Al fine di correggere tale errore, le parole «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione», devono leggersi: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione». Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

ringrazio, signor Presidente.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi è sconvocata. Per quanto riguarda la prossima settimana, avverto che in relazione ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge n. 1230, recante conversione in legge del decreto-legge sulla crisi dei mercati finanziari, la seduta antimeridiana di martedì 2 dicembre non avrà luogo. Resta inteso che nel corso di tale mattinata potranno proseguire i lavori di tutte le Commissioni. L'Assemblea del Senato tornerà a riunirsi martedì 2 dicembre, alle ore 17, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla crisi dei mercati finanziari. Ricordo che, come già comunicato ai Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento è stato fissato per le ore 12 di lunedì 1° dicembre. Avverto infine che la Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì prossimo alle ore 11, anziché alle ore 10 come precedentemente comunicato. **Per la

chi rimane in Aula rimanga con un minimo di tranquillità e di decoro. Consentiamo al senatore Perduca e agli altri iscritti a parlare di svolgere il loro intervento.

essendosi già presentata una simile situazione anche alla Camera nella scorsa legislatura, forse proprio per consentire l'istituzione della Commissione stessa e in vista della data del 10 dicembre, che è la Giornata mondiale per i diritti umani, si potrebbe chiedere a detto Gruppo di nominare il Capogruppo ed eventualmente procedere, una volta

Domani in Svizzera le varie organizzazioni di italiani residenti in quel Paese hanno organizzato, per questo *weekend*, una serie di manifestazioni e anche alcune occupazioni simboliche dei consolati di Losanna, San Gallo, Basilea e Zurigo. Nelle prossime settimane si svolgeranno ulteriori iniziative in altri Paesi. La motivazione è semplice. La finanziaria approvata alla Camera prevede un taglio di oltre il 50 per cento dei capitoli per le comunità di italiani all'estero. In modo particolare, ciò porterà alla chiusura dei corsi di lingua e cultura italiana, oggi seguiti da più di 600.000 ragazzi. Inoltre, il 7 dicembre prossimo si aprirà a Roma una prima Conferenza dei giovani italiani nel mondo. A questi giovani bisognerà che il Paese dia risposte se vuole costruire con loro

riguardanti l'introduzione del nuovo orario ferroviario a partire dal 14 dicembre. Vi sono delle problematiche chiare espresse in quella interrogazione, presentata da me, dal presidente emerito del Senato Marini e dal senatore Legnini, al ministro Matteoli e al ministro Tremonti. Ogni giorno io chiederò conto di questa interrogazione, perché è inaccettabile che il Parlamento non riceva risposte dall'Esecutivo su questioni importanti. Le Ferrovie potranno dire che non sono state attivate dall'Esecutivo proprio perché non c'è stata risposta del Governo. Se il metodo è quello di far passare il tempo in modo tale che la risposta non sia più necessaria perché superata

tenutasi in Commissione sanità della Regione Lazio, del rettore magnifico dell'Università di Roma, professor Luigi Frati, contestualmente anche preside della facoltà di medicina.

finestra")) che il direttore generale del Policlinico di RomaUmberto I, dottor Montaguti, non ha comunicato al preside della facoltà di medicina e al rettore magnifico la riduzione di 100 posti letto della prima e seconda facoltà di medicina,

tre studenti delle facoltà di medicina. La riduzione impone quindi una diminuzione degli studenti che possono partecipare ai corsi di medicina.

oltre ad essere presidente della Regione è assessore *ad interim* della sanità e commissario *ad acta* del Governo, quindi il taglio dei posti letto deve essere concordato con chi ne ha la responsabilità. Siamo preoccupati non tanto per i posti letto,

sul piano della sicurezza una categoria fra tutte è la più esposta, quella delle donne. Ad una donna come la signora Reggiani dovremmo dedicare, secondo me, non solo un ricordo, ma anche una riflessione approfondita su cosa intendiamo fare come istituzioni (oltre che come maggioranza e opposizione e come Governo), ma soprattutto come

La senatrice Bonfrisco ha posto un problema molto serio di impegno e di riflessione sui temi della sicurezza in generale